Onorevoli colleghi, cinque anni or sono, il Parlamento italiano consacrava la data di oggi, 10 febbraio, anniversario della firma del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate nel 1947, quale «Giorno del ricordo». Da allora, questa giornata è dedicata alla memoria delle migliaia di italiani dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia che, al termine del secondo conflitto mondiale, subirono indicibili violenze - quasi sempre per la sola colpa di appartenere al nostro popolo - trovando, molti di loro, una morte atroce nelle foibe del Carso. Quanti riuscirono a sottrarsi allo sterminio furono costretti a lasciare le loro case e ad intraprendere la via dolorosa dell'esilio: la popolazione italiana di quella regione fu quasi completamente sradicata, e fu così cancellata di colpo una presenza linguistica e culturale di tradizione millenaria, che traeva origine dagli insediamenti romani e si era consolidata con la Repubblica di Venezia. Su queste tragiche vicende calò per alcuni decenni, all'interno del dibattito pubblico del nostro Paese, un velo di omissione e di oblio, al punto che alcune voci autorevoli giunsero a denunciare la «congiura del silenzio», da parte della politica, della cultura e dei mezzi di informazione. Anche per effetto della celebrazione del «Giorno del ricordo», grandi progressi sono stati compiuti, in questi anni, verso l'obiettivo di una memoria matura e consapevole di tutti gli aspetti di quella dolorosa vicenda, affinché essa non fosse più motivo di scontro e divisione ma, al contrario, divenisse fattore di unità del popolo italiano, attraverso la celebrazione condivisa delle vittime di una tragedia comune. La legge che ha istituito il «Giorno del ricordo» si prefigge significativamente anche lo scopo di contribuire alla comprensione della storia complessa e drammatica della definizione del confine orientale del nostro Paese. Ed è proprio in quest'ottica più ampia e impegnativa che è necessario porre, a mio avviso, l'obiettivo di costruire una coscienza comune, tra i diversi Paesi della regione, e una memoria condivisa circa le cause e le responsabilità di quanto accadde in quegli anni. La storia europea degli ultimi decenni ci offre più di un motivo di conforto: l'avanzare del processo di integrazione europea ha consentito alle frontiere più chiuse di trasformarsi, in più occasioni, in confini segnati soltanto da cartelli stradali. Come è accaduto alla metà del secolo scorso con la frontiera franco-tedesca, così negli ultimi anni il progredire delle adesioni all'Unione europea ha consentito di compiere, anche nel quadrante orientale, i primi passi verso la ricucitura delle profonde ferite inferte dagli odi nazionali. La rimozione dei controlli di frontiera tra l'Italia e la Slovenia, a seguito dell'adesione di quel Paese all'Unione europea nel 2004, ha costituito una tappa essenziale di questo cammino, cammino, che ha visto anche i significativi risultati raggiunti dalla commissione storico-culturale italo-slovena, istituita nel 1993 per giungere ad una valutazione comune sulla questione delle foibe e sulla memoria di quell'eccidio. Alcune reazioni suscitate, in Paesi vicini, dalle parole che il Presidente della Repubblica ha pronunciato in occasione del «Giorno del ricordo» del 2007, dimostrano però, purtroppo, che rimane ancora molta strada da percorrere prima che si giunga ad una lettura comune degli eventi e delle responsabilità,

siano anche accompagnate da una pacata riflessione su quella dolorosa vicenda, in tutta la sua profondità storica. Un momento di riflessione che trovo particolarmente necessario in una giornata come quella odierna, in cui tutto il Paese è addolorato e commosso, qualunque fossero le opinioni individuali, per la conclusione tragica della vicenda di ieri, che costringe le nostre coscienze a confrontarsi con i temi della sofferenza, del dolore, della memoria, della dignità umana, della responsabilità. Per questi motivi e nel ricordo commosso di quanti patirono nel corpo e nello spirito l'atroce violenza delle foibe, invito tutta l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei che questo non fosse un momento uguale a tanti altri e

a chi di competenza perché venga stilato il semplice verbale di un momento in cui quest'Aula fa finta di occuparsi (come spesso e volentieri capita) dei problemi, mentre invece ha ben altro da fare. Spesso guardando alla mia sinistra mi accorgo come i rappresentanti della Lega sembrino essere i più titolati ad essere presenti, stipulanti e doverosamente attenti alle problematiche del Paese e e ai contenuti dell'incontro tra Presidente e senatori. Cosa dovrei dire? Che nel 1943 e nel 1945 Tito ed i suoi

del liceo classico Mele stanno facendo una grande manifestazione per non dimenticare la caccia all'italiano - scrivono loro - per ricordare Norma Cossetto,

Signor Presidente, ricordiamo oggi, per il quinto anno consecutivo, una delle più infami tragedie subite dal nostro popolo: la pulizia etnica con la sparizione e soppressione crudele di migliaia di nostri concittadini di ogni età, sesso e ruolo sociale, colpevoli solo di essere italiani. vicenda crudele come lo fu il forzato esodo dei nostri profughi e l'abbandono delle loro cose e della loro terra.

anche di molti altri italiani. All'epoca si scrisse, parlando del popolo dei profughi, «non riusciremo mai a considerare aventi diritto ad asilo coloro che si sono riversati nelle nostre grandi città non sotto la spinta del nemico incalzante, ma impauriti dall'alito di libertà che precedeva o coincideva con l'avanzata degli eserciti liberatori. I gerarchi, i briganti neri, i profittatori, che hanno trovato rifugio nelle città, che sperperano le ricchezze rapinate e forniscono reclute alla delinquenza comune non meritano davvero la nostra solidarietà né hanno diritto a rubarci pane e spazio che sono già così scarsi». Sono parole antiche,

La storia che noi oggi vogliamo ricordare è stata per tantissimi anni ignorata, ridimensionata e addirittura negata. Anche noi abbiamo avuto il nostro negazionismo. Ancora adesso esiste un rigurgito di negazionismo. Abbiamo recuperato alla nostra storia questa tragedia, ma non è ancora sufficiente. Serve una decisione più convinta, serve più condivisione, serve che questa pagina della nostra storia abbia l'adeguato risalto nella scuola e quindi nella formazione degli italiani. Serve - ed è un auspicio - che la tragedia delle foibe diventi una pagina della storia dell'Europa, condivisa da tutti gli europei o da coloro che vogliono ritenersi tali o che ritengono di sentirsi tali.

Proprio il 10 febbraio 2007 Giorgio Napolitano, il Capo dello Stato, disse: «Va ricordato l'imperdonabile orrore contro l'umanità costituito dalle foibe. (...) E va ricordata la "congiura del silenzio", la fase meno drammatica, ma ancor più amara e demoralizzante dell'oblio. Anche di quella non dobbiamo tacere, assumendoci la responsabilità dell'aver negato, o teso a ignorare, la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità politica, e dell'averla rimossa per calcoli diplomatici e convenienze internazionali». Mi auguro, signor Presidente, ed è un invito che rivolgo anche al Governo, che gli atti della commissione culturale italo-slovena

che ancora nel 2007 in un'Aula del Parlamento si è ritenuto non necessario che venissero resi pubblici in quanto già riconosciuti dalla parte slovena, ma non dalla parte italiana,

nel mondo della cultura e della scuola. Sarebbe un gesto concreto ed importante, che appartiene alla nostra storia. *(Applausi Signor Presidente, colleghi senatori, oggi celebriamo in quest'Aula il Giorno del ricordo che una legge del Parlamento nel marzo 2004 ha istituito per ricordare le vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e della più complessa vicenda del confine orientale, terre venete di millenaria tradizione. Sono stato uno dei promotori di questa iniziativa, perché per troppi anni si è ignorata una delle vicende più tristi e strazianti della nostra storia più recente, per troppo tempo dimenticata e ignorata, per non dire travisata. Fino al 1984 una cartina stradale edita da una delle più importanti case editrici del nostro Paese indicava le foibe come «grandi tombe piene di fascisti», un'offesa che è durata fino alla metà degli anni Novanta, quando cominciarono a trapelare i particolari, consentendo agli italiani di conoscere la verità storica di quel periodo. Fu un rigurgito di pura bestialità. Le foibe con la Resistenza non c'entrano, signor Presidente, ma sono il prodotto del comunismo staliniano. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. La ricerca della verità deve andare avanti, anche attribuendo responsabilità a chi allora occupava militarmente Trieste, americani ed inglesi, che fin dall'autunno 1944 ebbero notizia delle foibe ma preferirono non intervenire ma preferirono non intervenire per non irritare Tito, che consideravano un alleato sul fronte antinazista. Nel 1996 un magistrato di Roma,

italiano per l'inchiesta, tanto che il 15 giugno 1996, nell'aula del tribunale dove si svolgeva il processo, espresse il suo disappunto. «Mi chiedo» - disse Pititto - «perché lo Stato italiano per cinquant'anni non ha fatto questo processo, mi chiedo perché lo Stato italiano non sorregga il magistrato che in questo momento finalmente fa questo processo, mi chiedo perché la stampa italiana voglia mantenere il silenzio su questa che certamente è una vergogna per il nostro Paese». Era un chiaro atto d'accusa verso le istituzioni, che fino ad allora avevano pilotato gli eventi storici per paura di evocare episodi che potessero in qualche modo cambiare l'ordine della storia d'Italia. Quanta responsabilità in quel silenzio, quanta responsabilità in quanti hanno voluto occultare la verità, in quanti hanno voluto stravolgere la realtà per manipolare le coscienze collettive in favore di false ideologie. Una brutta pagina della storia italiana, poiché oltre a consumarsi un imperdonabile orrore contro l'umanità, si è attuata quella che il Presidente della Repubblica e lei lo ha citato, signor Presidente - ha voluto definire nel suo discorso di commemorazione del febbraio del 2007 con le parole del professor Barbi «la congiura del silenzio, la fase meno drammatica ma ancor più amara». Questa è una giornata per il ricordo di una storia negata, per il ricordo di una storia occultata che oggi più che mai è opportuno ricordare, anche e soprattutto per questo. Ragioni politiche, convenienze internazionali e ideologiche hanno relegato queste atrocità nell'ombra e nel silenzio. Oggi ed ogni anno in questo data, attraverso questo atto ufficiale, riconosciamo non solo il dolore ancora vivo nei famigliari degli infoibati, ma finalmente restituiamo dignità alle vittime, alle loro famiglie, alla stessa storia, facendo luce sulle responsabilità politiche. È ora che anche nei testi scolastici, signor Presidente, vengano ricordati con verità quei tristi avvenimenti e che finalmente i responsabili di quell'ingiustificabile silenzio vengano esplicitamente citati. Deve essere sconfitta l'ideologia che ha tentato di nascondere quello che accadde in quegli anni, anche con la ingiustificabile connivenza del comunismo italiano. Non dobbiamo dimenticare gli esuli fiumani, istriani e dalmati cacciati dal comunista Tito, diretta conseguenza della cultura dell'odio e della violenza che ha provocato i massacri delle foibe. Non possiamo dimenticare la posizione che i comunisti italiani assunsero in quegli anni: quella di contrastare gli esuli, costretti a lasciare tutti i loro beni e le loro case; e per quanto riguarda il risarcimento la ferita è ancora aperta, drammaticamente aperta e dovrà essere posta sul tavolo della trattativa per l'ingresso della Croazia nell'Unione europea. Pagine di storia così coperte di vergogna, signor Presidente, come quella che ricordiamo oggi, non devono essere dimenticate né cancellate e l'istituzione di questo Giorno del ricordo fa onore a tutti noi. *(Applausi dai Grazie, signori senatori, cinque anni fa una legge della nostra Repubblica, chiudendo un tempo lungo, troppo lungo, di silenzio colpevole, di rimozione, ha aperto una stagione nuova nella lettura di una parte significativa della storia del Novecento nel nostro Paese. Ha riportato al centro della nostra memoria collettiva il dramma di migliaia e migliaia di italiani istriani, fiumani e dalmati vittime delle foibe o costretti all'esodo dalla loro terra. La memoria. Per decenni, «foibe» è stata una parola presente nella nostra mente di italiani che non veniva mai pronunciata. c'era un'altra parola, «infoibati», tremenda nel suo significato e pessima nel suo stesso orrendo suono, che era stata anch'essa totalmente rimossa e cancellata dal nostro vocabolario: infoibati era una parola che in troppi avevano paura anche solo di pronunciare. Ma la memoria - è stato scritto - dà forma e senso alla vita, proteggendola dal nulla e dall'oblio. Con il Giorno del ricordo che oggi celebriamo, l'Italia ha iniziato un cammino, che forse sarà lungo, per uscire da quel nulla e dall'oblio e prendere finalmente coscienza di un passaggio drammatico e crudelissimo, ma incancellabile della sua storia. Oggi ricordiamo come al termine della Seconda guerra mondiale negli anni che sono seguiti, al confine orientale del nostro Paese, politiche di persecuzione giunte sino a forme di vera e propria pulizia etnica abbiano sconvolto un'intera, nobilissima e bellissima Regione, la Venezia Giulia. L'obiettivo tragico e, insieme, criminale di chi ha commesso il delitto delle foibe e di chi le ha volute era quello di annullare un popolo e, con la sua morte fisica, di distruggere la straordinaria esperienza culturale del popolo giuliano. Oggi, 10 febbraio, ricordiamo tutte le vittime di quegli anni, i morti, nonché le violenze, le prevaricazioni che nei luoghi occupati dagli iugoslavi vennero perpetrate dal regime comunista titoista contro la popolazione di quella terra già colpita dalle persecuzioni del ventennio fascista. E qui voglio anche ricordare, come uguale debito della memoria, il dolore e le persecuzioni subite dalla minoranza slovena durante il fascismo e durante la guerra. Nella tragedia, quelli delle foibe sono stati anche anni di sconfitta delle elevate tradizioni cosmopolite della città di Trieste e di tutta la Venezia Giulia, territori segnati da una formidabile dimensione multiculturale e dalla presenza sociale e culturale di consistenti e nobili comunità slovene e croate. È singolare, ma penso che non sia un caso, che la morte nelle foibe, le persecuzioni e la repressione abbiano colpito non solo i cittadini del Friuli-Venezia Giulia e gli abitanti di Trieste, Gorizia, Fiume e dell'Istria tutta, ma anche tanti italiani rimasti oltre il confine, vittime di un esilio massiccio e crudele. Dobbiamo alla volontà e alla forza degli italiani che vivevano fuori dalla loro Patria se, in un contesto storico e politico difficile e spesso ostile, sono stati mantenuti vivi

e nel lavoro contadino. Con il Giorno del ricordo, l'Italia ha iniziato un cammino, per uscire dal nulla e dall'oblio e prendere finalmente piena coscienza di un passaggio drammatico, crudelissimo, ma incancellabile, delle nostre vicende nazionali. Signor Presidente, stiamo parlando di una Regione italiana posta al centro dell'Unione europea, dove vivono tanti giovani. Ed è a loro, ai giovani del Friuli‑Venezia Giulia, che dobbiamo chiedere non solo di ricordare, ma anche di essere protagonisti di un vero processo di rinnovamento e di progresso, fondato sulla verità, sulla giustizia e sulla pace. E con questa celebrazione, oggi, nel giorno in cui si ricordano i martiri delle foibe, il Senato della Repubblica onora

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il Parlamento, istituendo il Giorno del ricordo, ha inteso riconciliare l'Italia con la sua storia e con quella grande tragedia che ricorda l'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati. Una giornata dedicata dallo Stato alla celebrazione ed alla memoria del martirio degli italiani infoibati, al loro assassinio di massa organizzato dalle bande partigiane e comuniste del maresciallo Tito, oggi considerato il primo raccapricciante segno di pulizia etnica attuata in quelle terre che durò fino al 1948 e provocò l'esilio forzato di 350.000 italiani, tra i quali vecchi, donne e bambini delle terre di Istria, di Fiume e di tutta la Dalmazia. Il Giorno del ricordo è un gesto di riconciliazione e di giustizia nei confronti di una pagina oscura e volutamente dimenticata per troppi anni che ha segnato la fine del Novecento. La finalità della legge n. 92 del 2004 è anche quella prevista dall'articolo 1, comma 2, cioè diffondere la conoscenza di quei tragici eventi, con particolare riferimento agli studenti di ogni ordine e grado; di svolgere una forte campagna di informazione storica e culturale; di sensibilizzare la conoscenza a 360 gradi di tristi eventi che hanno caratterizzato negativamente la storia del nostro Paese. Dall'entrata in vigore della legge, tale ricorrenza è stata celebrata da parte delle più alte cariche dello Stato e numerose iniziative sono state poste in essere da quasi tutti i partiti politici. Sono state altresì effettuate celebrazioni storiche, iniziative editoriali, trasmissioni televisive volte a rendere sempre più conosciute ai cittadini quelle tragiche vicende che, fino a marzo 2004, sono sempre state volutamente e colpevolmente dimenticate. Purtroppo non possiamo non denunciare, signor Presidente, che ancora oggi in Italia c'è chi intende minimizzare la tragedia delle foibe e che paradossalmente è proprio la scuola istituzionale a dimenticare maggiormente questa pagina tragica della nostra storia recente. Infatti, i testi di scuola dovrebbero contemplare questa tragica vicenda e, invece, in molti casi la stessa non viene nemmeno menzionata, disattendendo in questo modo una delle principali finalità della legge. della legge. Non si tratta semplicemente di disattendere la finalità della legge n. 92 del 2004, ma di proseguire volutamente in un processo di mistificazione e di falsità della nostra storia. Questo non permetterà il superamento dei rancori, degli odi, dei veleni che hanno così aspramente e negativamente caratterizzato le divisioni ideologiche nel nostro Paese, che anziché rimanere rilegate alla storia del fine Novecento, rischiano di indebolire il bisogno di una pacificazione nazionale rispetto ai tragici eventi legati al secondo conflitto mondiale. tenga presente che su 15 testi di storia analizzati, tra quelli in uso nelle scuole medie superiori, solamente cinque fanno menzione delle foibe. Per quanto riguarda i testi di storia adottati nel corrente anno scolastico nelle scuole medie superiori, numerosi non citano né le foibe né l'esodo. Desidero in questa occasione, signor Presidente, colleghi senatori, sensibilizzare ulteriormente il Governo per gli impegni assunti verso gli esuli in materia di risarcimenti relativamente ai loro beni, risarcimento che ammonta ad un miliardo di dollari. Voglio ricordare che il ministro Frattini si è già soffermato sul tema dei beni abbandonati anche in occasione della sua recente visita in Croazia. Il completamento del processo di riconciliazione e la definitiva integrazione sociale, culturale ed economica di Italia, Slovenia e Croazia sotto l'egida dell'Unione europea deve essere compiuto attraverso l'ascolto attento, l'interlocuzione ed il coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli esuli (in primo luogo, l'Unione degli Istriani), i quali sono ancora in attesa di un atto di giustizia, ancorché morale, che ne risarcisca il sacrificio pagato in nome e per conto dell'Italia uscita sconfitta dalla seconda guerra mondiale. Il 20 febbraio corrente Il 20 febbraio corrente mese al liceo scientifico Cavour di Roma avrà luogo una celebrazione per il Giorno del ricordo, alla quale parteciperà, oltre al professor Augusto Sinagra, ordinario di diritto europeo

Tutto questo, signor Presidente, fa parte di una corrente di pensiero negazionista? Possiamo tollerare che tanta disinformazione e falsità storica avvenga all'interno del sistema scolastico nazionale? Possiamo concepire che si continui a seminare odio e discriminazioni? Mettiamo al bando, con la forza della verità storica, ogni forma di negazionismo, se vogliamo far trionfare nel Paese e fra le future generazioni il principio di libertà e il rispetto dei diritti fondamentali ed inalienabili dell'uomo. Io penso - e mi avvio alla conclusione - che solamente ispirandoci ai valori della libertà responsabile, che si manifesta con il comportamento, noi potremmo svolgere un servizio al Paese nel rispetto delle nostre istituzioni e nel ricordo di quanti hanno sofferto e perso la loro vita non solo nelle foibe sul confine orientale, ma in tutti quei momenti atroci che hanno caratterizzato la fine del Novecento nel nostro Paese e in Europa. E per ricordare, signor Presidente, la congiura del silenzio, desidero ricordare solamente il nome di un caduto nella grande mattanza delle foibe. Vi finirono molti sacerdoti, ma, fra questi, don Angelo Tarticchio, che fece una fine simile a quella di Cristo: con una corona di spine fu crocifisso e poi infoibato.

intervenuti, con la celebrazione di questa giornata, istituita da un voto a larghissima maggioranza del Parlamento di alcuni anni fa, si compie anche un gesto di riconciliazione nazionale. Ed è importante, per il Paese, ritrovare sul proprio passato, sulla propria memoria, anche rispetto ad episodi tragici che sono appartenuti a pagine tristi della nostra storia e del nostro passato, un sentimento di unità nazionale. Solo a partire da un sentimento condiviso della storia, della memoria, del ricordo degli eventi più tragici del nostro Paese e delle zone di confine del nostro Paese,

Grazie,

Nel 1946 andò in Istria e venne a sapere delle foibe. Seppe di questo orrore terribile, di questo eccidio, di cui in quel momento al Sud non si sapeva niente, ne scrisse su «Rinascita». Scrisse un articolo sulle foibe su «Rinascita» ed ebbe, per questo, l'approvazione di Negarville, che era l'ideologo del Partito comunista. Qualche giorno dopo subì un processo interno, segreto, dal partito. Per questo fu sospeso per sei mesi dal Partito comunista; partito che, naturalmente, lasciò

così fortemente la libertà. Il negazionismo è cominciato nel 1946.

tutti gli interventi che si sono succeduti sono stati interessanti a vario titolo. Due questioni non sono state forse focalizzate. La prima è che, al di là del tempo trascorso dalla fine della guerra e dalla legge che ha istituito questa giornata,

cercato di dare una soluzione a due problematiche che, a sessant'anni di distanza, rimangono aperte, ossia la restituzione dei beni agli aventi diritto i risarcimenti, che finora sono stati dati con il contagocce dal Governo italiano, valutando i beni lasciati in Istria e in Dalmazia con parametri di valore del 1938.

causa anche - sottolineo la parola anche - della tragedia delle foibe e a causa di un clima di terrorismo instaurato in quelle terre, dovettero andare via lasciando tutto. Forse uno dei problemi è anche dovuto all'associazionismo degli esuli che, nelle sue espressioni più importanti (la Federazione degli esuli, l'Unione degli Istriani, l'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia), non è stato in grado sinora di indicare unitariamente ai vari Governi che si sono succeduti delle strade da percorrere. Ovviamente, i Governi che si sono succeduti ne hanno fatto tesoro: se non sapete voi quello che volete! Forse questi erano casi in cui il Governo italiano avrebbe dovuto dire che cosa proponeva.

Su questo tema c'è sempre stata molta sordità da tutte le parti.

In entrambi non emerge dal quadro complessivo degli interventi una singola misura dalla quale si possa dire con certezza che sarà di stimolo al rilancio dell'economia. Non c'è una linea politica di sostegno al reddito che possa funzionare da stimolo ai consumi; non c'è un sostegno sociale al problema più grave, che colpisce un tessuto sociale che diventa sempre più fragile.

il dato più preoccupante è quello della cassa integrazione straordinaria, che presenta una dinamica pari al 20,7 per cento. Come è noto, se la cassa integrazione ordinaria richiede un provvedimento dal carattere temporalein quanto conserva un'aspettativa di vita lavorativa, la cassa integrazione straordinaria si usa per crisi ormai irreversibili. Hovoluto fare questa premessa per sottolineare che bisogna tenere ben presenti i dati e guardare la realtà per quella che è e non per quella che a volte è comodo presentare con gli effetti di annunci prima fatti e poi smentiti. Allora,nel cosiddetto decreto milleproroghe si introducono nuovi ed ulteriori elementi di criticità. Innanzi la prassi che fa assurgere a forma ordinaria l'adozione di questo modello di decreto accresce, in una situazione già confusa, l'incertezza degli operatori dei diversi settori in vista di continui e sistematici rinvii.

31 dicembre 2010 l'efficacia delle disposizioni legislative in tema di IRAP e tassa automobilistica. non si fa altro che prolungare di ulteriori due anni normative emanate dalle Regioni in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, evidenziando che la deducibilità dell'IRAP stabilita dal cosiddetto decreto anticrisi non è altro che un piccolo rimedio ad una situazione di tassazione anomala, mentre resta il problema della stessa esistenza dell'IRAP, della base imponibile su cui si applica e delle complicazioni contabili che comporta; dall'altro lato, viene definitivamente posto nel dimenticatoio l'impegno elettorale del presidente Berlusconi di cancellare le tasse automobilistiche. Penso, inoltre, all'articolo 32 del provvedimento che proroga al 16 maggio 2009 i termini di applicazione sia della norma relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno

abbiamo il primato scandalo delle morti bianche e, secondo l'INAIL, vi sono 200.000 casi di infortuni non denunciati. Un rapporto dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro sottolinea che, a distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha stabilito nuove norme in materia di sicurezza sul lavoro, i coordinamenti provinciali delle attività ispettive stanno appena muovendo i primi passi, mentre il personale impegnato

disomogeneità, - mi riferisco alla mancata soppressione di enti inutili - fino a proroghe di strumenti che rinviano a norme non graditeal Governo, come l'articolo 19 sulle azioni collettive risarcitorie. Nella manovra dell'estate scorsa, approvata in Parlamento, l'articolo 26 recava il titolo altisonante "taglia enti" e prometteva di sopprimere, a sentire roboanti annunci dei ministri Brunetta e Calderoli, tutti gli organismi pubblici al di sotto dei 50 dipendenti:

si è scoperto che i ministri Brunetta e Calderoli avevano individuato solo nove enti che rientravano nei criteri della loro legge e, dopo un attento esame, li hanno confermati tutti e nove. Così, il "taglia enti" si è trasformato in un "salva enti" da potenzialmente inutili ad indispensabili o quasi, almeno per il momento. Basta pensare che una vera mappa ufficiale sul loro reale numero a tutt'oggi non esiste, un vuoto che rende quasi complice il susseguirsi dei rinvii. Ultimo della serie in ordine cronologico è proprio quello deciso dal Governo nell'ambito del decreto-legge milleproroghe per far slittare il termine per il ridimensionamento di quelli che possono definirsi veri e propri derivati tossici della burocrazia italiana. Parliamo di una lista, per una migliore comprensione dei colleghi, che secondo il cosiddetto elenco ISTAT, fino ad oggi preso a riferimento per lo sfoltimento di questi enti, comprende oltre 340 strutture. Se a ciò si aggiunge poi il capitolo dei comitati e delle commissioni ministeriali, l'ultimo censimento, portato a termine proprio due anni fa dall'allora ministro Santagata, parla di oltre 700 organismi individuati. Nel decreto-legge milleproroghe, inoltre, il Governo scopre le carte sulla *class action*. In Italia se ne discute da anni. Il Governo Prodi nel 2007 aveva tolto ogni incertezza introducendo nella legge finanziaria, mettendo in campo un serio tentativo di creare un sistema di protezione a tutela dei consumatori. È bene ricordare che all'epoca la reazione della Confindustria, dell'associazione delle banche e di quella delle assicurazioni era stata violenta. La *class action* era stata definita un attacco al sistema industriale italiano e così la volontà di modificare il testo ha già imposto due rinvii.

Restano poi forti dubbi sulla sostanziale esclusione della retroattività, tanto da rendere impossibile a tanti risparmiatori vittime dei *crack* di questi anni ottenere risarcimenti a ristoro delle perdite subite. Che dire poi della politica

poi l'articolo 41, comma 16, rinvia gli effetti della riforma fino al 30 giugno 2009. In pratica, resta tutto com'era. Le amministrazioni avranno sei mesi in più per assumere i lavoratori a termine con i criteri dettati dal Dipartimento della funzione pubblica e se l'amministrazione non potrà farlo subito potrà comunque prorogare il contratto a termine, cosa che invece nella precedente formulazione

andrebbe bene se il provvedimento fosse, come lui accennava, anticrisi o di carattere strutturale riguardo all'economia e al fisco. Ciò non è.

ampie, precise e specifiche ragioni e, se vogliamo, giustificazioni. Per esempio, ricordare la proroga dell'entrata in vigore della *class action*

per renderla strumento utile al cittadino e non potenzialmente dirompente rispetto alla realtà delle imprese o degli enti pubblici. Oltretutto si dice nella relazione che si spera di cambiarla in tempi brevi senza aspettare il 30 giugno 2009, dando così la possibilità agli uffici giudiziari di attrezzarsi rispetto a questo nuovo strumento giuridico che, come tutti sappiamo, essendo uno strumento giuridico rivoluzionario per la realtà del nostro Paese,

è profeti a caso se si pensa che quando entrerà in vigore la *class action* i primi mesi saranno di assalto alle sedi giudiziarie, perché ognuno avrà qualche contenzioso da porre in essere o al quale aggregarsi. Pertanto, la nostra giustizia, già così gravata, si troverà in serissima difficoltà. responsabilità di tutti noi arrivare a migliorare questa norma e prepararsi a renderla diritto vivente nel nostro ordinamento e nel nostro sistema sociale. sociale. Non voglio soffermarmi sulle critiche del collega e neanche

che risulterebbe inutile per le ragioni che ho detto, essendo l'analisi del testo già stata ampiamente sviluppata, e per iscritto e oralmente. Vorrei far invece notare e ricordare

il presidente Vizzini ed il relatore Malan in prima linea, insieme ai sottosegretari Giorgetti e Casero.

socialità, intesa sotto diversi profili, non solo quello delle imprese e degli enti pubblici, ma anche altri, riguardanti momenti importanti dell'applicazione della nostra Costituzione.

fra quelli del Governo, intendo ricordare, perché ne parleremo nelle prossime ore,

riguardante disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie.

l'inasprimento delle pene o giri di vite esagerati. Il diritto alla sicurezza e l'esercizio dei poteri in materia di sicurezza

guardiamo alla nostra realtà carceraria e consideriamo come ormai il numero di detenuti sia almeno doppio rispetto a quello di coloro che possono essere ospitati negli istituti di pena, che l'indulto si è dimostrato un provvedimento che non ha svuotato le carceri, se non per pochi mesi, che le condizioni dei carcerati sono pessime, sono pessime, comprendiamo tutta una serie di fenomeni che ci occupano in Parlamento e sui *mass media*.

buonsenso del giudice ed al suo buon diritto e non alle valutazioni improvvisate di chi non conosce il caso), occorre anche ricordare come l'ingresso di un giovane in carcere finisce per diventare per lui non solo un momento particolare di afflizione

Abbiamo una Carta costituzionale che non dobbiamo mai dimenticare (quanto ne abbiamo parlato nelle scorse, tragiche ore) che all'articolo 27 (lo ricordo per me) recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Possiamo

- non ne parliamo - ai fini rieducativi dei condannati. Infatti, a fianco di fortunati istituti carcerari ove c'è il lavoro interno e addirittura si consente un lavoro esterno controllato,

"cessi", chiamiamoli pure così, alla turca per evitare che i topi salgano su e vengano a far visita ai detenuti, di tantissimi scarafaggi che circolano insieme ad altri animaletti in queste celle umide, invivibili, caldissime d'estate e freddissime d'inverno. Quando, ogni tanto, pensiamo ai carceri turchi, ai carceri tailandesi non guardiamo la nostra realtà

voi sapete che chi entra in cella, soprattutto se è giovane, spesso subisce violenze sessuali, veri e propri strupri, che non avrà mai il coraggio di

che non succeda più. Dobbiamo allora ringraziare il Governo e, primo fra tutti, il ministro Alfano quando interviene con questa norma per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri. E comunque fino al 31 dicembre 2010 al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti poteri speciali al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire - sottolineo - una migliore condizione di vita ai detenuti.

facendone un ente dotato di personalità giuridica con la possibilità di finanziare, tra l'altro, progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie con procedure snelle che la Cassa delle ammende attuale si sogna. Queste sono cose che andavano fatte da anni; sappiamo la sorte dei denari che che arrivano alla Cassa delle ammende, sappiamo anche la sorte dei tantissimi denari che non vengono incassati per la lentezza di una particolare burocrazia. Si spera di riuscire, attraverso questo meccanismi agile, a portare a casa tutto il dovuto e nel contempo a mettere a disposizione

alla collocazione in edifici non strettamente carcerari, della quale si è parlato diffusamente a livello di enti locali per persone di minore pericolosità. Presidente e colleghi, ho fatto l'esempio

*(IdV)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, naturalmente noi diamo un giudizio molto severo su questo decreto che rappresenta l'ennesima e sistematica utilizzazione di uno strumento normativo, per sua natura temporanea, a fini di aggiustamento e correzione della legislazione in vigore mediante varie forme di modulazione di termini e di scadenze. Il decreto di proroga termini sembra ormai divenuto una tipologia a sé stante, un oggetto di per sé omogeneo in base al quale confrontare le singole disposizioni. Ci si inventa in tale modo un nuovo parametro ormai scontato, mentre non sono scontate le conseguenze di un simile atteggiamento. La prassi dell'adozione sistematica di questo tipo di decreti-legge non può che determinare un giudizio - ripeto - severo e negativo, soprattutto perché da parte del Governo si dimostra un atteggiamento che conferma l'inclinazione a considerare tale tipologia normativa come una forma ordinaria d'intervento del Parlamento stravolgendo letteralmente i principi e gli equilibri contenuti nella Carta costituzionale. Non voglio ripetere ciò che é stato già detto anche da altri colleghi, soprattutto dal senatore Mascitelli, Mascitelli, sul rinvio alle calende greche, ancora per una volta, di uno strumento di tutela dell'azione collettiva da parte dei cittadini, che doveva entrare in vigore Il senatore che mi ha preceduto ha affermato che ci sarebbe un assalto alle sedi giudiziarie

sotto diretta dettatura di banche, assicurazioni e Confindustria; voglio ricordare, infatti, che ci sono 450.000 risparmiatori frodati dai *bond* argentini, 145.000 dal *crack* della Parmalat, 35.000 da Cirio, che abbiamo il problema della Lehman Brothers, il problema di altre frodi e truffe finanziarie, la portabilità dei mutui che, nonostante la legge Bersani, non è stata applicata dalle banche e pertanto non accade nulla. Voglio ricordare l'anatocismo bancario, ossia la prassi delle banche di derogare a precise norme del codice civile Grazie, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la commissione di massimo scoperto, ossia quello che è stato definito un pizzo legalizzato, che è stato dichiarato illegittimo ed illecito dalla Cassazione, viene ancora praticato. Non si venga a dire che è stato sanato perché qualcuno ha affermato nell'altro ramo del Parlamento che i cittadini... *(Brusìo)*.

Grazie, signor Presidente, stavo affrontando il problema, magari per chi non voleva ascoltare, dell'azione di classe, ossia uno strumento di tutela per i diritti dei cittadini, che era stato faticosamente approvato un anno e mezzo fa e che doveva entrare in vigore. Ripeto, questo strumento non va, come ha detto il collega che mi ha preceduto, ad intasare le aule giudiziarie, ma semplifica snellisce le procedure, dà una possibilità ai frodati ai truffati. È anche un strumento di deterrenza, perché le imprese le imprese serie che vogliono stare sul mercato non hanno nulla da temere. Anche questo è stato rinviato alle calende greche, a data da destinarsi e i cittadini, i consumatori, soprattutto in una fase come questa, di grave difficoltà economica, ancora privi di un importante strumento di tutela. Sorvolo sulle altre questioni che riguardano questo provvedimento, come ad esempio il taglio agli enti pubblici non economici, l'adeguamento IRAP e tasse automobilistiche regionali, i concorsi pubblici riservati, la questione dell'ISTAT, il pagamento delle sanzioni irrogate dall'Antitrust. Ma voi forse ce l'avete proprio con l'*Antitrust*, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato: prima la volete depotenziare e poi addirittura, in un momento come questo, per attenuare gli effetti della grave crisi economica in atto, prorogate di trenta giorni il termine per il pagamento delle multe irrogate dall'Antitrust nell'anno 2008. Sorvolo sul contrasto al terrorismo internazionale: per aprire esercizi pubblici di telefonia ed Internet adesso è obbligatorio, anche per tutto il 2009, la licenza da richiedere al questore. Ci sono poi altre questioni che riguardano il Codice delle assicurazioni, la proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, la proroga di termini in materia di accantonamento, la liquidazione coatta amministrativa dei concorsi agrari, e

signori rappresentanti e onorevoli colleghi, questo articolo è una vera e propria liberalizzazione delle molestie telefoniche. Quando i dati personali presenti nelle banche dati, costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005, sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costruire dette banche dati prima dell'agosto 2005 (ossia la norma del garante per la *privacy*) vuol dire che voi liberalizzate le molestie telefoniche. Le famiglie,

tra le altre liberalizzazioni, anche quella delle molestie telefoniche. Mi auguro che ci sia un ripensamento da parte della Commissione, mi auguro che possiate tornare indietro. Vedete, ci sono tante questioni che attengono ad una crisi economica dura, che viene dagli Stati Uniti, al fatto che magari le manovre anticrisi non sono adeguate, al fatto che le piccole e medie imprese non ce la fanno più, al fatto che le famiglie devono tirare la cinghia e non ce la fanno più a far quadrare il loro magro bilancio, ma se a tutto questo aggiungete anche la liberalizzazione delle molestie telefoniche, voi portate la responsabilità di inserire all'interno della pace famigliare molestie che potrebbero essere evitate. *(Applausi dal

il provvedimento di cui discutiamo concerne la conversione in legge del decreto-legge n. 207 del 2008, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

sono particolarmente sottolineate alcune questioni relative al mantenimento ed alla garanzia dei livelli di sicurezza nel nostro Paese. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 11 del provvedimento,

Credo che questa sia una misura assolutamente importante, necessaria per mantenere alta la vigilanza sui pericoli che incombono

misura, tuttavia, pur incanalata nell'alveo del potere legislativo dello Stato alla stregua dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione,

deve tenere conto che, in funzione ed in ragione della legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha modificato il Titolo V della Costituzione, in materia di polizia amministrativa vige un riparto di legislazione concorrente con le Regioni. prima della riforma costituzionale del 2001, ricordo che la legge Bassanini, con il decreto legislativo n. 112 del 1998, aveva assegnato questa potestà legislativa diretta a prevenire e limitare danni e pregiudizi per i cittadini, ciò che compendia l'attività autorizzatoria delle pubbliche amministrazioni, appunto, alla polizia amministrativa, in quanto tale alla potestà legislativa concorrente con le Regioni. Ora, sappiamo che l'esercizio della potestà legislativa concorrente tra Stato e Regione concerne l'individuazione dei criteri da parte dello Stato, mentre la legislazione di dettaglio è delegata alle Assemblee legislative regionali. Non v'è dubbio che il contrasto al terrorismo internazionale sia una specifica materia di competenza dello Stato; ciò nondimeno, questo tipo di attività deve essere svolta coinvolgendo anche i livelli e le potestà degli enti autarchici territoriali cui la nostra Costituzione conferisce un potere legislativo, appunto Sono quindi convinto che questa norma non debba avere un carattere transitorio (il decreto-legge la proroga fino alla fine dell'anno 2009), ma che debba essere incardinato un regime permanente, pur con le differenziazioni di cui testé

che tratta delle disposizioni in materia di ricostruzione dei debiti degli imprenditori agricoli della Regione Sardegna:

fuori? È una mancanza di rispetto per chi interviene. complesso, costituito dal fatto che una decina d'anni fa una legge aveva consentito a migliaia di imprenditori della Regione Sardegna di accedere a forme di credito agevolato.

degli imprenditori agricoli di adempiere a queste obbligazioni. Ora, sappiamo che nella materia dell'agricoltura la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni è limitata,

proprio perché queste esigenze si radicano nel più complesso diritto di tutti i cittadini italiani alla tutela della proprietà privata e del diritto di impresa. del Parlamento, anche ieri abbiamo discusso a lungo sui principi fondanti e fondamentali della Costituzione repubblicana. Credo però che accanto ai diritti di libertà, così come li conosciamo e sono sottolineati, non vi sia dubbio alcuno che la proprietà privata ed il diritto di impresa siano assolutamente intangibili e connessi alla libertà personale. il senatore Pera sottolineava appunto come tra i diritti inalienabili della persona umana che si radicano nell'articolo 2 vi sia il diritto alla vita, alla libertà personale, a tutto ciò che il giusnaturalismo, sin da Thomas Hobbes, nel 1500, aveva individuato nel contrattualismo costituzionale di livello europeo. Ebbene, il diritto di proprietà rappresenta nel modo più assoluto e fondamentale l'esplicazione di questi diritti. Sappiamo persino che nell'ambito della costruzione dell'Unione europea, quindi nel primo pilastro, il diritto dei trattati, ma anche nella costruzione delle delle politiche agricole che riguardano la cooperazione e la costruzione del complesso edificio dell'Unione europea, perfino richiamato dal Trattato di Lisbona, c'è un intervento anche da parte delle Regioni, un intervento significativo, posto che il sistema europeo è un sistema federale che riconosce le autonomie territoriali degli Stati, le autonomie che noi conosciamo a livello regionale. senza pensare a procedimenti di infrazione di fronte alla Corte di giustizia europea e debba anzi, senza infingimenti, con la massima determinazione, avviare

L'ultima considerazione, signor Presidente, la voglio indirizzare al problema dell'edilizia penitenziaria. Si tratta di un problema di grande civiltà. Qui ci siamo battuti per introdurre delle norme severissime, in particolar modo per l'introduzione di procedimenti direttissimi. Pur tuttavia sappiamo che metà della popolazione carceraria del nostro Paese è costituita da cittadini extracomunitari e, quindi, è urgentissimo garantire a chi subisce limitazioni della libertà personale il rispetto di quella dignità e quelle condizioni carcerarie che fanno del nostro Paese uno dei Paesi più avanzati. In fondo, replicando a quel che diceva il collega Boscetto, c'è da sottolineare che in nessun Paese del mondo e in nessun Paese liberale occidentale c'è stato un giurista come Beccaria, che aveva sottolineato la tutela della dignità umana. Nel 1789 negli Stati Uniti d'America,

inoltre al giudice di affidarglielo perché attraverso il lavoro lo avrebbe rieducato. Nel 1789 negli Stati Uniti si introdusse il *probation*, cioè la libertà condizionata per il reinserimento sociale. Pensate, nel nostro Paese, queste argomentazioni sulla civiltà del diritto - perché il diritto non è mai affermazione dell'autoritarismo dello Stato, ma riconoscimento dei diritti - già c'erano John Probation traeva l'istituto del *probation*, quindi della libertà vigilata, dall'opera di Cesare Beccaria, il quale era stato portato negli Stati Uniti da un mecenate fiorentino che aveva scritto, insieme a Thomas Jefferson, la Costituzione degli Stati Uniti e che si chiamava Filippo Mazzei. Quindi, vedete come, nel contesto internazionale dei delitti e delle pene, l'Italia,

italiani è quello della solidarietà, della fraternità, del perdono e della rieducazione di chi ha sbagliato. Quindi, anche queste misure sull'edilizia carceraria sono misure che noi adottiamo e approviamo. Nei mesi precedenti, infatti, abbiamo aggravato le sanzioni per i responsabili di alcuni reati; ma, attraverso queste misure di edilizia penitenziaria, sottolineiamo il grado di civiltà del nostro Paese e, soprattutto, l'intendimento di questo Governo di avviare

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché questa mattina ho ascoltato l'intervento del collega della Lega Rizzi. Vorrei attirare l'attenzione del Governo sull'effetto devastante e sul vero contenuto dell'emendamento che ha illustrato il collega Rizzi. Questa mattina egli ci ha presentato come una buona idea l'utilizzo dei fondi della legge n. 147 del 1997, da mettere a disposizione delle Province e dei Comuni penso della zona frontaliera.

i periodi di disoccupazione dei lavoratori frontalieri. È stato detto questa mattina dal collega Rizzi che, dal 1º giugno, la Svizzera pagherà direttamente gli indennizzi di disoccupazione, in seguito agli accordi bilaterali con l'Unione europea. europea. Così non è. Oggi la legge n. 147, alimentata - ripeto - non dalle casse italiane, ma dal lavoro e dalle trattenute sugli stipendi dei lavoratori frontalieri, prevede un indennizzo del 50 per cento dell'ultimo salario per 12 mesi. Dal 1° giugno di quest'anno, con gli accordi tra la Svizzera e l'Unione europea, la Svizzera verserà ai lavoratori frontalieri disoccupati

(il Governo dell'epoca) non ha trattato correttamente. Vorrei ricordare al Governo che gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea prevedono la possibilità di correggere correggere errori di questo tipo in trattati bilaterali. Sarebbe pertanto opportuno che il nostro Governo intervenisse nei confronti della Svizzera per rivedere l'applicazione di questo accordo. Ciò che però è assolutamente inaccettabile è presentare questo come un intervento nell'interesse dei Comuni e delle Province di quella Regione,

crisi. State attenti con il populismo e con il vostro modo di affrontare i problemi. Questi sono cittadini italiani, nel mio modo di vedere le cose; ma credo che, anche nel vostro delirio, sono cittadini padani, perché vivono su quel territorio. Vorrei attirare l'attenzione del Governo inoltre segnalare al Capogruppo della Lega, che questa mattina si è offeso per il fatto che un organo di stampa importante del nostro Paese ha definito leggi razziali alcune oscenità che la Lega ha imposto a questa maggioranza

che è stato sostenuto in un ordine del giorno che la Commissione ha accolto, e ciò mi sembra un po' superficiale da parte della Commissione. Vorrei attirare l'attenzione sul fatto che c'è anche un altro emendamento, che ho presentato.

e di lasciare questi fondi a disposizione per l'utilizzo per il quale sono stati creati e per versare i contributi di questa cassa di disoccupazione ai lavoratori frontalieri. Desidero altresì ricordare che, nell'ultima legislatura, i sindacati dei frontalieri vennero in Senato ad incontrare il Comitato per le questioni degli italiani all'estero e già all'epoca avevano segnalato il problema del cambiamento di regime e dell'utilizzo di tali fondi. Dunque, il mio intervento non vuole essere altro che un appello al Governo per evitare che si cada in questa

di stabilità; norme per garantire la vigilanza parlamentare sugli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; vi sono varie altre misure riguardanti diversi settori.

della completa affidabilità da parte degli uffici a questo preposti e, dall'altra, crea la concorrenza tra coloro che producono solo pezzi di ricambio rispetto a coloro che producono sia i pezzi di ricambio sia il veicolo originario.

delle prestazioni collegate al reddito per l'erogazione delle medesime. Dall'anno scorso si richiedeva ai percettori di una pensione di fare una dichiarazione per l'anno in corso

un contenzioso di decine di migliaia di casi con spese da parte del contribuente e da parte dell'ente previdenziale ed

Sono stati approvati interventi importanti con l'accordo di maggioranza e opposizione per quanto riguarda i fabbricati rurali: l'intento di evitare l'elusione fiscale facendo passare per rurale ciò che non è

tra quelli che forniscono un reddito a chi li possiede. Vi sono altri interventi di aggiustamento, ma credo che nel complesso sia stato svolto un lavoro positivo. Torno

Presidente, il confronto intorno al decreto-legge cosiddetto milleproroghe o proroga termini è un confronto che, dal punto di vista del metodo, si ripete ogni anno

situazioni relative alla pubblica amministrazione o di norme che non sono state del tutto rispettate o di adempimenti che dovevano essere chiusi entro le scadenze previste per legge in realtà necessitano di ulteriori proroghe.

che il Governo vuole ribadire, sostanzialmente legate a tempistiche di provvedimenti che necessitano di interventi di proroga, a questioni che rivestono priorità strategica per il Paese e che quindi, giustamente, le forze politiche possono decidere

che probabilmente invece tali questioni meritano. Pertanto, all'interno del provvedimento, come è stato ben ricordato dal relatore Malan, che ringrazio in questa sede per il lavoro svolto,

dando la disponibilità a valutare alcune di tali questioni e ad approfondirle. Quindi, signor Presidente, soddisfatto del lavoro svolto per quello che compete al Governo, anch'io mi associo ai ringraziamenti nei confronti

al quale sono stati presentati oltre 400 emendamenti. Pertanto, tenuto conto del lavoro svolto in Commissione, il Governo presenta un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge

in attesa che il Governo completasse le sue cose, vale a dire il maxiemendamento di cui ha parlato il ministro Vito. Sappiamo perfettamente che il Governo